Signor Presidente, la sensazione che si ha di fronte a questo provvedimento riguardante le modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli è quella di ritenere che, ultimamente, lo sport preferito praticato dall'attuale maggioranza di Governo sia quello di sgretolare, mattone dopo mattone, i pilastri su cui si fonda lo Stato italiano e la nostra convivenza civile. Non si programmano interventi strutturali a favore dell'economia, si dimentica frettolosamente che le famiglie hanno il solito problema irrisolto, nonostante il cambio di maggioranza, con la quarta settimana del mese, ma non sfugge all'intransigente azione del Governo che, tra le emergenze del Paese, spicchi prioritariamente la modifica degli articoli del codice civile relativi al cognome della moglie e dei figli. Con un atto apparentemente semplice, che si configura in linea con gli impegni cui reclama il Consiglio d'Europa e la Convenzione su ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, si intendono cambiare i princìpi che fanno parte non da oggi, ma da una tradizione millenaria che risale al diritto romano e che coinvolge l'assetto stesso della famiglia. Al di là del merito della questione, che può anche apparire suscitata da riscontri positivi, riguardanti sia i princìpi dell'ordinamento e del valore costituzionale sull'uguaglianza tra uomo e donna, sia nella discriminazione per i figli nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti dal padre, quello che desta non poche preoccupazioni è il tentativo di innovare radicalmente, di cancellare una tradizione - e le tradizioni appartengono ad un popolo - senza che la problematica relativa sia stata adeguatamente approfondita e dibattuta nel Paese, senza cioè che sia comparsa, muovendosi dalla società, una spinta, verso la modifica così come proposta. Preoccupa al riguardo come l'introduzione del criterio della variabilità, nel trasferimento del cognome, mutevole - o del padre o della madre o di entrambi con ordine concordato o persino alfabetico rischi di far perdere la riconosciuta continuità e la memoria tra le generazioni. La preoccupazione di introdurre tale modifica al fine di garantire - è detto - maggior rispetto dei diritti di entrambi i coniugi oltre che per contribuire ad una migliore integrazione della cittadinanza europea adeguandosi agli altri Paesi dell'Unione, ci sembra non fortemente rilevante. Compare nella relazione la comparazione, a proposito del principio di uguaglianza tra marito e moglie nella trasmissione del cognome dei figli, con varie legislazioni straniere, ma sfuggono dal ricordo i motivi che legano le questioni del cognome alla storia di questo nostro Paese e che in forma estremamente semplicistica vengono rubricate ad un mero residuo di società patriarcale. Ma così non è. Non so se abbiate percezione che ciò che emerge nella pubblica opinione è un profondo senso di perplessità e smarrimento verso una innovazione proposta e non richiesta e che si configura piuttosto fumosa nella sua attuazione. Nella relazione al disegno di legge si fa riferimento alla sentenza del 12 febbraio 2006, n. 61, della Corte costituzionale la quale afferma: «L'attuale sistema di attribuzione del cognome dei figli è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». Ora, se il punto di partenza viene configurato in una questione di raggiungimento dell'uguaglianza dei sessi o di affermazione di parità tra marito e moglie, sicuramente esso non può ritenersi superato se con il provvedimento che si intende adottare la scelta del cognome diventa un fatto meramente casuale. Infatti, pur prescindendo dalle complicazioni anagrafiche che l'attribuzione di due cognomi determina, c'è il rischio nemmeno tanto remoto che si ottenga l'effetto di attenuare i legami familiari piuttosto che consolidarli; di incidere sul principio di unità della famiglia che il legislatore costituente aveva inteso garantire, con la conseguenza che la famiglia non sia più considerata un soggetto collettivo, un'entità diversa dalle singole persone, ma diventi un insieme fin troppo casuale di soggetti. Stando così le cose, riteniamo sia davvero più urgente e proficuo che il Parlamento dia priorità ai temi della tutela, delle politiche adeguate, della condizione economica di una gran parte delle famiglie italiane, le quali non chiedono elemosine ma sostegni veri e concreti; che si diano cioè risposte alle nuove urgenze e alle sollecitazioni della storia; risposte prioritarie quindi alla famiglia con i suoi bisogni: la casa, innanzitutto, e poi il lavoro, sia quello che manca che quello precario. Riteniamo che questo provvedimento si muova nel solco già aperto dai DICO. Esso continua a navigare nella confusione ideologica, non piccola, che stenta ancora a riconoscere la maggioranza del nostro Paese, una maggioranza silenziosa, ma non sempre, così come testimoniato dal *Family Day*, una maggioranza che però saprà essere rumorosa in ogni circostanza in cui sono messi in gioco i princìpi su cui si fonda la nostra civiltà. Prima di mettere mano a modifiche del codice civile, sarebbe più opportuno approfondire il tema coinvolgendo in un ampio dibattito l'opinione pubblica e le organizzazioni che la rappresentano. Quest'Assemblea e il nostro Paese hanno questioni ben più importanti con le quali misurarsi e di certo le modifiche al codice civile in materia di cognome del coniuge e dei figli non ne rappresentano la priorità.

chi sta intervenendo ha avuto già modo di affrontare la tematica oggi all'esame dell'Aula nel corso della XIV legislatura, allorquando, congiuntamente, la Commissione speciale infanzia e minori e la Commissione giustizia affrontarono

arenarsi e morire di morte propria, sulla base di due semplici considerazioni. La prima è già riecheggiata ripetutamente nelle osservazioni e riflessioni sottoposte all'Assemblea dai colleghi che mi hanno preceduto, ovverosia l'assoluta indifferenza del corpo sociale rispetto a questo provvedimento; l'altra, che ancora forse non è stata adeguatamente sottoposta all'attenzione del Senato, ovverosia gli altissimi costi di impianto di tale riforma. Va detto infatti, ed è bene che tutti i colleghi lo sappiano, che, a prescindere da tutte le altre osservazioni e considerazioni già svolte, proprio nel corso di quel lungo e approfondito in costante contatto con i funzionari del Ministero dell'interno che si occupano degli uffici Anagrafe, si cercò anche di comprendere quali sarebbero stati i costi effettivi di siffatta riforma, venendo informati che gli stessi assommavano, nella migliore delle ipotesi, a centinaia di milioni di euro, solo per mettere in condizione gli uffici Anagrafe di poter recepire siffatta modifica. Credo che da queste due premesse si debba necessariamente prendere lo spunto per comprendere la sostanziale inutilità di ciò che stiamo facendo. In primo luogo, ripeto, vi è nel corpo sociale una totale indifferenza rispetto a questo provvedimento, non vi è alcuna espressa richiesta, anzi, opportunamente la collega Monacelli che mi ha preceduto ha ricordato come in campo familiare ben altre siano le esigenze. Del resto, mi chiedo e vi chiedo, onorevoli colleghi, quale sia la ragione, in assenza assoluta di segnali in tal senso provenienti dalla società italiana, di andare a incidere su una tra le più consolidate tradizioni della nostra gente, una tradizione che affonda le proprie radici non nei secoli ma nei millenni. millenni. È sufficiente ricordare che lo stesso termine patria, tanto caro a tutti noi, significa appunto terra dei padri

che di generazione in generazione si tramandano. Ciascuno le sente non soltanto come un'eredità di chi lo ha preceduto, ma come un patrimonio proprio da lasciare ai figli.

alla storia del nostro Paese; mi chiedo cosa potrebbero dire gli eredi di Giuseppe Garibaldi, di Giuseppe Mazzini, di Giosuè Carducci al pensiero che un semplice bisticcio o un semplice capriccio possano portare alla scomparsa di quei cognomi che sono stampati e che non appartengono soltanto a chi li porta ma alla storia di tutti noi. Se anche volessimo prescindere da tutto questo e volessimo ritenere che le tradizioni non hanno più un senso e un significato, anche sotto il profilo della semplice convenzione e della praticità del sistema non potremmo che pervenire ad identica ed analoga conclusione. Siccome non basta soltanto aspetto, ma è bene forse comprenderlo, mi sono preso - onorevoli colleghi, mi perdonerete se vi tedierò per un istante con una sorta di grottesca sciarada la briga di verificare cosa potrebbe accadere laddove si andasse ad impiantare questa legge, così come viene proposta. Cominciamo (non ha importanza se sia uomo o donna, perché di fatto siamo in un'assoluta reversibilità di posizioni) dal signor Bianchi che sposa la signora Rossi e il signor Neri che sposa la signora Azzurri (prescindo da ogni riferimento calcistico, che per quanto mi riguarda è scontato). I signori Bianchi-Rossi decidono di attribuire al proprio figlio il cognome Rossi; i signori Neri-Azzurri li attribuiscono tutti e due. Il signor Rossi, figlio di Bianchi-Rossi (e Bianchi è già scomparso), conosce la signorina Neri-Azzurri e decidono di sposarsi. A quel punto, di comune accordo espungono il cognome Neri e il cognome Rossi e si limitano a quello Azzurri. quello Azzurri. I loro figli si chiameranno soltanto Azzurri. In due semplici passaggi abbiamo già perduto tre cognomi, che non sono soltanto un dato anagrafico, ma sono la storia delle famiglie da centinaia di anni. Andiamo avanti. Il signor Azzurri, che sarebbe erede di Bianchi, di Rossi e di Neri, che ormai sono cancellati dalla storia di quella famiglia, conosce la signorina Verdi-Marroni. siccome questo è un mondo in cui ogni tanto le femminucce riescono a dirla più dei maschietti, l'unico cognome che viene attribuito è Marroni e quindi al terzo passaggio di cognomi ne abbiamo persi già cinque. Il signor Marroni conosce poi la signorina Gialli e anche in questo caso - ma non cambierebbe nulla se attribuissero il cognome Marroni - decidono di attribuirne uno solo. Che sia Gialli o Marroni ha scarso significato e tanto meno ne ha cromatico,

È questa la riforma che stiamo proponendo alle famiglie italiane, che ben altro ci chiedono? È di questo che siamo chiamati oggi a discutere, onorevoli colleghi: di una sorta di infernale e grottesca sciarada anagrafica, che la società italiana non ci chiede, che le è assolutamente estranea e che comporta costi di impianto altissimi, nell'ordine di centinaia di milioni di euro, non attestati dai parlamentari dell'opposizione, ma certificati dal Ministero dell'interno. La famiglia italiana ben altre cose ci chiede e vi chiede, non certamente questo. Nella Nella consapevolezza, tra l'altro già emersa nel corso dei nostri lavori, che il provvedimento, proprio per come è costruito, dovrà comunque tornare in Commissione, facciamolo semmai tornare in Commissione e cerchiamo di riesaminarlo attentamente alla luce di queste considerazioni, invece di costruire una sorta di ineffabile pastrocchio anagrafico solo sulla base di un progressismo di maniera che ritenevamo avesse finalmente fatto il suo tempo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, intervento affermando con estrema sincerità che tutto mi sarei aspettato di discutere, in questo tempo della XV legislatura, meno che un disegno di legge per le modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli. In Senato non stiamo discutendo e approvando che pochissimi disegni di legge; per lo più, portate alla nostra attenzione ratifiche di decreti-legge o leggi di delega al Governo. Anche fra le forze della maggioranza sono esplose polemiche roventi in proposito, polemiche che hanno prodotto l'intervento dello stesso Presidente della Repubblica. Avete ridotto ad un terzo l'attività legislativa delle Camere rispetto a quanto accadeva cinque anni fa, durante il Governo di quelle che con disprezzo e arroganza definite le destre. Ebbene, quelle destre - come dite voi, senatori della maggioranza - avevano dato o tentato di dare risposte vere alle mille urgenze del Paese. Voi, con incredibile superficialità, di fronte a molte difficoltà e ritardi della pubblica amministrazione e dello Stato, rispetto alle esigenze del Paese, proponete la riforma del cognome. Sono centinaia i disegni di legge che l'opposizione ha presentato; segno evidente di una nostra grande capacità di analisi e di proposta, segno che vogliamo essere fedeli al buonsenso e al dovere di responsabilità verso i nostri concittadini. Di tutti i disegni di legge presentati finora fate emergere dopo mesi questa vostra sul cognome, frutto non del buonsenso, ma di evidenti esigenze ideologiche che hanno trovato spazio nel vostro fumoso e contraddittorio programma. Certamente era nel vostro programma e i programmi elettorali vanno rispettati, ma un po' di logica e di opportunità politica potevano consigliarvi di preferire altri provvedimenti a questo. Non sto discutendo della legittimità della proposta; ogni disegno di legge deve poter trovare spazio in quest'Aula. Ciò non significa tuttavia che non debba e non possa essere giudicato da un punto di vista etico o, al limite, della sola opportunità politica. Mi domando: c'è una vera esigenza di questa legge? Quali problemi andrebbe a risolvere? Quale vera spinta sociale muove questo provvedimento? Quali questioni di natura giuridica già emerse andrebbe a regolamentare? Nessuna di queste domande trova adeguata risposta sia nel testo della legge, sia nella relazione che vorrebbe motivarla. Non ci sono questioni giuridiche serie da normare, normare, problemi da risolvere; non c'è una spinta sociale evidente - questa è la cosa più importante - neanche promossa da una minoranza un po' significativa. Non c'è, in sostanza, nessuna vera esigenza perché questo provvedimento venga adottato. Forse è solo un'esigenza ideologica della maggioranza; non vorrei, tuttavia, che più che un'esigenza diventasse una sorta di capriccio. Nella relazione si citano, come di consueto, le legislazioni di alcuni Paesi europei, le raccomandazioni del solito Consiglio d'Europa e di qualche altra istituzione, ma non c'è un'analisi seria del nostro Paese. Credo sia arrivata l'ora di vincere questo quasi inguaribile provincialismo italiano che deve motivare le proprie scelte sempre guardando ad altre esperienze. Perché la relazione non prende in seria considerazione l'analisi della società italiana, cercando lì le eventuali motivazioni? Come valuteranno, ad esempio, il milione e oltre di partecipanti al *Family day* un simile provvedimento? Certamente le poche migliaia presenti a Piazza Navona l'avranno considerato necessario o addirittura urgente. Voglio rispettare il pensiero di quella piccola piazza, ma credo che il Parlamento debba guardare con altrettanto rispetto - se non superiore, almeno per il numero che esprimeva - il sentimento e l'idea della sterminata e stracolma Piazza San Giovanni del 12 maggio scorso. All'inizio della relazione si dice che l'attuale normativa non garantisce che ciascuno sia se stesso anche nel cognome che porta e che si debba garantire un'effettiva pari dignità ad entrambi i genitori nei confronti dei figli. Parole grosse, colleghi senatori; parole grosse per giustificare un piccolo provvedimento; parole al limite del ridicolo, se debbo veramente pensare che un giovane, un uomo o una donna del nostro Paese, debba sentirsi veramente se stesso perché ha un cognome diverso. diverso. La crisi di identità dei nostri giovani è maturata per ragioni completamente diverse dal loro cognome paterno. Forse, proprio la demolizione della figura del padre ha prodotto in molti giovani, soprattutto maschi, la difficoltà a crescere, a trovare il giusto equilibrio e la necessaria sicurezza per affrontare con coraggio e responsabilità le scelte che la vita impone. Molti autori hanno scritto della cosiddetta eclissi del padre e forse dovremmo preoccuparci di questa più che di altro. La figura del «padre *bancomat*» risulta sempre più prevalente e anche il nostro sistema scolastico lamenta l'assenza della figura del maestro, a tutto vantaggio delle insegnanti donne. della fine della leva obbligatoria è venuto meno un altro tipo di educatore maschio, così come sono praticamente scomparsi gli educatori d'oratorio, che pure sono stati fondamentali nella nostra educazione di ragazzi in preparazione del ruolo di padre, e questo indipendentemente dai nostri convincimenti ideologici e, forse, anche religiosi. Quelle che sto facendo sono delle semplici constatazioni, evidenti a tutti, vere perché appartenenti alla nostra esperienza. Per questa ragione, è paradossale affermare che il disegno di legge miri a garantire che ciascuno sia se stesso anche nel cognome che porta. L'affermazione è paradossale e la legge finisce per essere contraddittoria rispetto ad essa, laddove afferma - appunto - che essere se stessi dovrebbe essere garantito da una scelta di cognome. Quale sarebbe, infatti, la differenza fra la trasmissione del cognome paterno e una possibilità di scelta con quello materno, oppure con entrambi o ancora con una successione alfabetica dei cognomi dei genitori? Un essere umano sarebbe più se stesso con il cognome della madre o con quello di entrambi? Portando a logica esasperazione il principio che la legge vuole affermare, un individuo sarebbe se stesso solo battezzandosi in proprio e scegliendo il proprio nome e cognome, come accade in America con le targhe delle automobili. Ma come è possibile sapere chi si è se non si conosce l'altro? E se si spegne la conoscenza dell'altra persona più importante della mia vita, dell'altro che mi ha dato la vita e mi ha generato, come si può sperare di diventare qualcuno?

Queste le domande che ci sono rivolte fin da piccoli. Con ciò, non avendo comunque il cognome della propria madre nella carta d'identità, non ci siamo sentiti meno persone, né meno noi stessi. Pertanto, non con questa motivazione, ma semplicemente unendo al cognome paterno quello della madre daremo corso legislativo ad una prassi largamente condivisa senza retoriche ideologiche, senza inutili femminismi di maniera, senza scomodare gravi riconoscimenti di uguaglianze sociali negate a danno delle nostre madri. Nessuno di noi ha mai avuto bisogno di chiamarsi con il cognome materno per

Comunque, è l'altra motivazione di fondo della relazione introduttiva a suscitare ulteriore e benevola ilarità. Arrivare ad affermare che l'effettiva pari dignità di entrambi i genitori nei confronti dei figli garantita dalla scelta del cognome fatta di comune accordo o, in assenza di accordo, fatta con la casualità dell'ordine alfabetico non può che suscitare un certo umorismo. Credo che la pari dignità debba essere misurata e valutata in ordine alla responsabilità educativa, alla volontà effettiva di costruire una famiglia che protegga e faccia crescere in serenità i figli; forse, anche in ordine all'affetto, alla dedizione, alla capacità di testimoniare sacrificio, senso del dovere, partecipazione alle cose buone; forse anche in ordine all'amore vero e disinteressato che un genitore è capace di donare. Credo che nessuno di noi abbia avvertito la propria mamma in una sorta di diminuita dignità, perché non dava il proprio cognome alla prole: credo che ciascuno di noi abbia misurato la dignità del proprio padre e della propria madre solo in relazione al bene di cui erano capaci e non ad una fredda ed oggettiva condivisione o condizione nominalistica stabilita per legge. Questa legge non serve, se non nella limitata parte nella quale aggiungerebbe a quello paterno il cognome materno. Ci sono infatti questioni di natura pratica che mi sembra non prendiate in considerazione; questioni di natura organizzativa ed anche economica, che andrebbero a pesare enormemente sui nostri Comuni. Abbiamo altre emergenze: abbiamo molte altre cose sulle quali concentrare le nostre energie e le nostre attenzioni. Il dibattito sulla famiglia, per esempio, invece che a Firenze sotto campagna elettorale, l'avremmo potuto fare da subito in quest'Aula, viste le già numerose proposte di legge presentate sull'argomento; invece no: siamo costretti a parlare di DICO e di modifica della disciplina sui cognomi. Queste sarebbero le grandi conquiste di civiltà e di uguaglianza sociale delle quali il Governo e la maggioranza sono capaci. Non è un caso che vi allontaniate sempre di più dal sentire comune; non è un caso che questo Governo registri i più bassi indici di gradimento mai verificati per un Esecutivo nel nostro Paese. Se questi indici altamente negativi fossero il frutto di scelte coraggiose, impopolari ma necessarie, sarei il primo a darvene atto. Non sono preconcettualmente contrario a tutto ciò che proponete. Proprio di recente, e per ben due disegni di legge delega al Governo, ho dichiarato il voto positivo dell'UDC. La nostra, lo ribadiamo, è un'opposizione responsabile e coscienziosa, che valuta le cose e valuta le soluzioni proposte. Qui, per questo caso, valutiamo che il vostro distacco dal popolo italiano è abissale, perché vi preoccupate di questioni inutili e marginali e non avete il coraggio di affrontare la realtà che attende altre risposte. Se la vostra impopolarità fosse maturata intorno a questioni e risposte serie, forse l'UDC sarebbe insieme a voi a condividerla; se, per esempio, aveste affrontato in modo serio, onesto ed adeguato l'ordinaria gestione dei rifiuti in Campania, contro le demagogie ambientaliste e gli interessi malavitosi, non avrei potuto non dichiarare il mio apprezzamento. Invece, anche lì, solo chiacchiere e fumo negli occhi: purtroppo, questa volta, il fumo delle centinaia di mucchi di rifiuti che vengono incendiati per disperazione da popolazioni fin troppo pazienti. Cosa dicono, in proposito, certi grandi giornali nazionali di Bassolino e del sindaco Iervolino, gli stessi che salutavano il loro ingresso al potere in Campania e a Napoli come una sorta di svolta messianica, che ha avrebbe finalmente dato civiltà e certezza del diritto ad un'area del Paese distrutta dal sottosviluppo e dal malgoverno? Era il grande modello per lo sviluppo del Sud, secondo la ricetta della sinistra. Perché nessuno di questi giornali oggi tira in ballo e intervista il presidente della Regione Campania? Sono troppo occupati a parlare di DICO, di doppio cognome e a travisare la realtà della manifestazione di Piazza San Giovanni. Di questo dovremmo parlare seriamente. Credo, cari senatori della maggioranza, che avete sbagliato bersaglio, ma siete in tempo per rimediare. Questa vostra proposta è tutta fuori campo, perché tra l'altro va ad indebolire ulteriormente proprio quella figura - il padre - che andrebbe invece sostenuta e rivalutata. Su questi argomenti non si può scherzare. Per stare all'amato provincialismo, un piccolo studio comparato delle legislazioni esistenti in questo settore in Europa ci dice che anche l'avanzatissimo Nord-Europa, tanto attento ai diritti delle donne, non è arrivato a simili incredibili proposte. Una legge può anche essere sbagliata, perché non risponde nel modo migliore ad un bisogno reale: questo tipo di legge è la norma in ogni ordinamento; ma un ordinamento legislativo che introduce norme inutili e praticamente non richieste tradisce il suo stesso fine: servire il popolo e non le idee di pochi. Per questo credo che, con un adeguato atto di coraggio, la maggioranza in quest'Aula, o una parte di essa, potrebbe salvarci da questo disegno di legge; basterebbe un po' di onestà intellettuale per farlo, riconoscendo questa proposta come non urgente. Noi non grideremmo alla vittoria, ma semplicemente riconosceremmo il prevalere del buon senso nei partiti di Governo. Nella cosiddetta Prima Repubblica accadeva normalmente che su un disegno di legge anche importante si ritornasse più volte fosse accantonato per lungo tempo e ripreso dopo importanti ed adeguate modifiche. Con ciò non cadevano Governi, né si gridava alla lesa maestà del potere della maggioranza, che magari superava largamente il sessanta per cento e non come ora che sopravvive con uno scarto di frazione d'unità; semplicemente prevaleva la saggezza e l'arte parlamentare consigliava percorsi più morbidi rispetto agli scontri e alle barricate. Mi permetto di consigliarvi un medesimo comportamento. È scandaloso - dico e ripeto: scandaloso - che la risposta al *Family day*, all'emergenza sociale delle nuove famiglie povere, alla mancanza di dignità (questa sì vera e fondata sulla mancanza di lavoro, di risparmio, di disponibilità economica minima, ma anche di protezione sociale, di nuove emergenze sociali che colpiscono i giovani nelle nostre famiglie), si risponda con questa amena e poco significativa proposta; non è il momento per farla, prima risolviamo i veri problemi della famiglia e poi occupiamoci dei ricametti giuridici sui cognomi. Questa visione della coppia e della famiglia è vecchia e reale, nessuno può essere veramente interessato al doppio cognome se non una ristretta *élite* borghese ed illuminista. Una coppia giovane che vuole sposarsi, di tutto sente l'esigenza meno che del doppio cognome: vuole un lavoro stabile, vuole poter acquistare una casa a prezzi accessibili, vuole attenzione fiscale dallo Stato e dai Comuni; credo non voglia più assistenza come se fosse una emergenza sociale da combattere e risolvere. La famiglia è un soggetto che, assumendosi un'enorme complesso di doveri, reclama semplicemente diritti: non diritti a danno di altri e contro qualcuno, diritti per poter agire e compiere in libertà quelle scelte necessarie per essere se stessa. Vogliamo e vogliono che la famiglia possa essere se stessa: questa è la richiesta della grande maggioranza delle famiglie, le stesse che con il 75 per cento di non voto hanno bocciato il *referendum* contro la legge n. 40, le stesse che a centinaia di migliaia hanno manifestato la loro gioia di essere unite con molti bambini, portando la testimonianza di una Italia che non viene mai rappresentata dai *media*; eppure è un'Italia che esiste, che cresce, che offre speranza al Paese, che non picchia i poliziotti, che non pretende nulla senza prima aver dato e che riceve sempre meno di ciò che ha offerto al Paese. Chiediamo ai milioni di giovani che intendono sposarsi o comunque avere dei figli, se preferiscono una legge sul cognome o una finanziaria che destini ogni anno qualche miliardo di euro in più alla famiglia. Liberiamo la famiglia dall'oppressione fiscale che questo Governo ha imposto, diamo alla donna madre la dignità economica, riconoscendo con interventi concreti il suo lavoro e la sua funzione sociale, magari con consistenti sgravi fiscali per ogni figlio che ha messo al mondo e che sta faticosamente crescendo rinunciando a qualsiasi altra carriera nel lavoro e nella società. Vado alla conclusione, signor Presidente. Questa è la vera uguaglianza sociale: riconoscere la libertà della scelta della donna e dell'uomo che vogliono diventare genitori. Per i figli che nascono il vero problema non sarà il cognome che sarà ricevuto, ma la serenità dei loro genitori nel crescerli. Questo è oggettivamente un bene e compito dello Stato è anche quello di riconoscere il bene dei cittadini e mettere questo al di sopra d'ogni altro. Ho forti dubbi che i cittadini italiani riconoscano la riforma del cognome come un vero bene; credo piuttosto che serva ad alimentare il clima di sfiducia e disinteresse verso la politica quando questa è lontana dalle vere esigenze di bene e felicità. Il dibattito in corso potrà non essere del tutto vano se sarà servito a farvi riflettere e ripensare a questa proposta: è il nostro appello al buon senso che ci auguriamo possa prevalere nei banchi della maggioranza.

abbastanza semplice; fuori del Palazzo ci sono circa 60 milioni di italiani che oggi si pongono soltanto la domanda: ma dentro i Palazzi sono tutti impazziti?

pensionistico previdenziale. È proprio di questi giorni il punto dell'efficienza del sistema politico e dei costi della politica;

Ebbene, a 60 milioni di italiani che vi chiedono una cosa voi rispondete: vi daremo una legge che cambierà il metodo con cui attribuire il cognome ai coniugi e ai figli.

Oggi si vive in un modo un po'diverso, più concentrati in grandi scatoloni di cemento e a volte anche i postini hanno difficoltà a trovare i recapiti dei destinatari della corrispondenza. Pensiamo cosa accadrebbe se questo sciagurato disegno di legge entrasse in vigore: un postino si rivolge al

Fallito nella storia, si ripercorre come progetto politico molto più raffinato ad ogni piè sospinto.

sistemi, un parlamentare è espressione ed ha mandato di un corpo elettorale e prova a tutelare gli interessi,

in questo ambito o in quest'altro, di cambiare sistema per attribuire cognome ai figli? Forse viviamo in un posto fuori dal mondo, in mezzo ai barbari, incivile; noi sentiamo la gente che ci chiede: infrastrutture, meno tasse, più lavoro, più occupazione

ma qui c'è uno scardinamento dell'uno e anche dell'altro. Chi parla vi dice come la pensa, ma non crede di essere così avulso dal mondo: io amerei continuare a potermi chiamare come si chiamava mio nonno, almeno so da che parte sono arrivato, non come una meteora su questo pianeta, amerei che i miei figli e i miei nipoti potessero ricordarsi di me se non altro perché portano il mio cognome; così è stato, così ci siamo abituati, senza stravolgere i modi di vita di nessuno, senza toccare i diritti degli uomini e delle donne, crediamo sia un modo normale di poter vivere. Un monito Un monito a questa sinistra: perché ci si prende la libertà di stravolgere il modo di interpretare le relazioni tra le persone? Questa è una grande arroganza. Perché ci si prende la libertà di distruggere un modello sociale che è il modello della famiglia, come a piè sospinto continuate a fare? Chi vi dà questa libertà? La libertà

salvo poi indignarsi se qualcuno ironizza su altre religioni, perché quelle sono intoccabili: la laicità vige e le offese si possono fare soltanto nei confronti della religione interna. Guardate, anche l'ostentare le diversità dove esiste una grande tolleranza in questo Paese non è una cosa così normale; per il *Gay Pride* in Russia, dove c'è un tradizionalismo ortodosso canonico che non si scuote: non erano *naziskin*, quelli che hanno picchiato i vostri parlamentari, io li ho visti, erano donne, erano nonne, che tiravano bottiglie perché dicevano: «Noi tolleriamo anche il modo di vivere dei diversi, ma non venite qua ad ostentarlo come per dire che bisogna cambiare i valori della nostra società. Cacciateli, tornate in Italia, se lì vi si consente, da noi queste cose non sono consentite». C'è anche una carenza di libertà, è vero, c'è una carenza di espressione di libertà e di espressione democratica, ma c'è una grande volontà di mantenere le tradizioni, volontà che voi avete, purtroppo, perso in questo Paese. Vi porto un piccolo particolare, che deve servire a far capire come a volte le tradizioni riescono a imporsi sull'evoluzione dei diritti.

esiste l'antica Regola feudale di Predazzo: si tratta di proprietà collettive che danno diritto ai partecipanti di usufruire

l'avente diritto è la famiglia con determinati requisiti che trasmette il diritto in discendenza verticale maschile. discendenza verticale maschile. Il genitore che non mette al mondo maschi fa perdere il diritto ai discendenti. È giusto? È sbagliato? È così dal 1500.

non sono diritti indisponibili della persona, ha ritenuto più forte il diritto tradizionale che non quella sbavatura sotto il profilo dell'uguaglianza, che non consente alle donne di beneficiare alla stessa maniera della parte maschile. Questo per dire quanto le tradizioni nel nostro Paese sono ancora rispettate e lo sono al punto che a volte possono anche forzare i diritti moderni. Desidero dire una cosa alla maggioranza: potete fare ciò che volete, potete fare le leggi che volete, potete indebitare il Paese fin che volete (d'altronde avete voi le chiavi della cassaforte); vi chiediamo però una cosa: non stravolgete il nostro modo di vivere, ciò che è stato fino ad oggi.

fatto parlare di distacco dalla politica, distacco dalla politica che c'è stato da parte degli elettori di sinistra nei confronti dei loro riferimenti politici e che una certa campagna di stampa ha cercato di definire come fenomeno generale,

con articoli quotidiani su certi giornali ben schierati e ben orientati, seguiti magari da una discesina in campo di qualche importante esponente dell'antipolitica che dalla politica ha ricevuto ogni sorta di benefici. Non c'è stato nulla di tutto questo, eppure stiamo discutendo dei cognomi. Tuttavia, non dirò che questo non è un provvedimento importante. È un provvedimento importante, anzi lo è anche troppo. Come è stato già detto, su questioni del genere che riguardano la famiglia non viene prima la legge e poi la cosa: viene prima la cosa, la consuetudine, la tradizione che la legge cristallizza, che la legge norma e ne fa una regola applicabile nei casi di incertezza. È talmente vero questo che - ad esempio - per quanto riguarda l'attribuzione ai nuovi nati

un bambino o bambina venga attribuito il cognome del padre. Non c'è scritto da nessuna parte: questo fatto è determinato dalla consuetudine, dalla tradizione talmente forte che le eccezioni - quelle sì - vengono normate dalla legge. Vorrei ricordare che ci vuole molta prudenza prima di intervenire su una materia di tal genere. In tutti i Paesi è vero questo. I Paesi che sono intervenuti per forza di legge a modificare una consuetudine generalmente non sono stati Governi particolarmente democratici che avevano a cuore la libertà. A nessuno è venuto in mente di modificare - per esempio - la tradizione islandese dove non esiste un cognome ma solo il patronimico. L'islandese, oltre al nome suo proprio che gli viene attribuito dai genitori, ha non il cognome di famiglia ma il nome del padre - naturalmente il nome proprio del padre

proprio. Nel nostro Paese, l'ultima volta che si è intervenuti con forma di obbligo sui cognomi, è stato un intervento, che non mi risulta di legge, per l'italianizzazione di certi nomi, per cui - grazie al cielo - solo in alcuni casi e non in modo sistematico i Wiesenthal del Südtirol sono diventati Vallebianca

però, devo dire che quel Governo non è ricordato per il suo libertarismo e tantomeno per essere stato *politically correct*, perché era il regime fascista. se si interviene su una materia di questo genere, ritengo si debba essere molto attenti e credo che, se davvero si ritiene di intervenire, occorra farlo rispettando due cose fondamentali: la libertà e la consuetudine. Fino ad oggi è successo, come ho detto, senza neppure che questo fosse scritto in alcun testo di legge, che nessuno sceglieva il cognome dei figli visto che era dato dalla consuetudine, per cui automaticamente al bambino veniva attribuito il cognome

per quanto riguarda il cognome dei figli - nulla dovrebbe cambiare nell'attribuzione del cognome stesso e dovrebbe continuare ad essere attribuito il cognome del padre. Invece, se c'è una espressa volontà da parte di entrambi i genitori di attribuire il cognome in modo diverso, ad esempio, come è già scritto nell'attuale testo di legge approvato dalla Commissione è la possibilità di avere entrambi i cognomi con in primo luogo il cognome del padre e poi quello della madre o viceversa, oppure solo il cognome del padre, oppure solo il cognome della madre, credo che, anche alla luce di quanto è stato detto dalla Corte costituzionale - la quale però ha precisato che tocca al legislatore fare scelte in questo senso, che saremmo noi mi ricorda opportunamente il Presidente della Commissione giustizia - toccherebbe a noi certamente intervenire ma, naturalmente, con discernimento perché altrimenti significherebbe scrivere leggi sotto dettatura. Vi sono anche delle decisioni di organismi internazionali che però - lo ricordo - non hanno impedito, ad esempio, alla Spagna, che ha sempre avuto la tradizione del doppio cognome, cioè del cognome del padre seguito da quello della madre, di mantenere la tradizione ove non ci fosse una scelta di consenso da parte dei genitori, per cui adesso, in Spagna, è possibile mettere per primo il cognome della madre e solo per secondo il cognome del padre ma, in caso di mancata decisione, resta per primo

Ci possono essere delle necessità o ci può essere semplicemente la libera scelta da parte dei genitori di imporre il doppio cognome o il cognome della madre. In Germania si può fare, anzi, in Germania addirittura è possibile che che il marito assuma il cognome della moglie, e conosco qualcuno che ha fatto questa scelta. Se è una scelta libera, perché no? Inoltre, ci sono anche queste decisioni della Corte costituzionale, ma non può essere imposto come obbligo, e dobbiamo anche essere molto attenti nel porlo come opportunità perché è evidente che tale possibilità di scelta può generare litigi, può generare malanimo fra le famiglie dei genitori che si contendono il primo posto, o l'unico posto nella graduatoria. Dunque, nei casi ove venga richiesto e si ritenga di fare altre scelte, credo potremmo esaminare questa possibilità, ma imporla come obbligo - e vedo che ci sono parecchi emendamenti e disegni di legge in questo senso - è veramente indice di un cattivo modo di riferirsi alla società da parte del legislatore: il fatto di voler cambiare la

Allora, credo che dobbiamo essere veramente molto cauti in questo tipo di leggi. E aggiungo un punto:

Può sembrare una esigenza, questa, che va in direzione di una migliore tutela della donna. Sono del parere che, ove ci fosse un consenso da parte dei genitori, questo può sicuramente essere fatto. Ma non dimentichiamo che c'è anche un altro tipo di evoluzione nella nostra società. Non vi è soltanto un ruolo della donna, non paragonabile certamente a quello della donna di cento, ma anche di è una parità dal punto di vista della legge assoluta. Vi sono delle difficoltà in alcuni settori, l'abbiamo dibattuto anche riguardo alla

non soltanto dei figli nati fuori dal matrimonio da coppie di fatto, ma dei figli abbandonati, ignorati dai genitori e, particolarmente, dal padre. Il fatto che avvenga più spesso che il padre si disinteressi dei figli piuttosto che la madre, è evidente; anche questo è - ahimè! - tradizionale; ma privare il padre di questo legame obbligatorio nei confronti dei figli può in qualche caso voler dire giustificare il colpevole il colpevole disinteresse che a volte arriva al punto di non partecipare, come è preciso dovere dei padri, al sostentamento dei figli. Non è una mia

in certi aspetti di estremismo, sia nelle concrete conquiste che hanno avuto, una delle quali si sta manifestando, senza alcun obbligo di legge in questi mesi, in cui uno dei principali, forse il principale candidato alla Presidenza è proprio una donna, e non perché è una donna, ma perché è ritenuta da moltissimi elettori la persona più adatta a ricoprire quella posizione. Ebbene, l'argomento portato da numerose femministe molto attente in quel Paese è stato proprio quello: di fronte ad un numero sempre maggiore di padri, che si disinteressa dei figli o al limite che si interessa dei figli solo per quanto sono obbligati dalla legge, cioè nel mantenimento meramente economico e non all'educazione, alla presenza, che è dovere di un padre oltre che naturalmente di una madre (ma in questo secondo caso le inadempienze sono più rare o meno evidenti), proprio in nome di questo, molte femministe si sono dette che non serve questo provvedimento, anzi rischia di andare verso un'ulteriore deresponsabilizzazione dei padri, specialmente quando i figli nascono fuori dal matrimonio, e dunque al di fuori di un legame che obbliga che obbliga anche nei confronti del coniuge e non soltanto naturalmente nei confronti dei figli. Ci sono dei punti importanti di questo provvedimento che vanno comunque esaminati io ritengo con attenzione, anche ove si decidesse di soprassedere - cosa che non mi rattristerebbe particolarmente - alla normativa sui cognomi, come quello riguardante completa parificazione dei figli per quanto riguarda i diritti, senza distinzione tra i figli nati all'interno del matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio. Questo è un punto molto importante e

Nella nostra società si ritiene unanimemente che i genitori abbiano degli obblighi e un legame nei confronti dei figli del tutto indipendente dalla condizione

di creare problemi dove invece si vogliano risolvere. Quanto al resto, torno a ripetere che, prima di intervenire su un istituto talmente forte che non è neppure stabilito dalla legge ma unicamente dalla consuetudine, con la forza sua propria, occorre fare molta attenzione. Non è importante in questi casi la velocità. A volte sembra che il Parlamento debba essere giudicato in base alla velocità, ma credo sia la qualità il requisito fondamentale di ogni nuova legge. Se per la qualità è necessaria qualche settimana in più di dibattito o un ritorno in Commissione, credo che sicuramente la stessa vada privilegiata, specie in questo settore dove, accanto a

Ove ci sia piena libertà di scelta, sono del parere - ho anche presentato un emendamento in questo senso - che si possa pensare di applicare il provvedimento non soltanto ai nuovi nati che non abbiano fratelli maggiori della stessa coppia,

Uno degli aspetti del matrimonio, o comunque dell'unione di due persone per generare figli, che produce particolare coesione sociale è la mobilità sociale da matrimonio, ovvero il matrimonio tra persone di strati sociali diversi.

tendenza ancora più ridotta da parte di famiglie con cognomi altisonanti, in particolare da parte dei maschi, a prendersi una moglie con un cognome meno illustre e meno altisonante, per evitare che i propri figli abbiano un cognome che sia un ossimoro sociale, cioè con un primo cognome di particolare rilievo e prestigio e un secondo cognome più popolano. Naturalmente, l'auspicio di tutti è che si scelga la propria moglie e il proprio marito secondo altri criteri, ma non possiamo negare la realtà. Si potrebbero fare anche alcuni esempi di

inglese, i primi principi nella linea di successione, il principe Carlo, il principe William e suo fratello, devono il proprio ruolo alla loro nonna e non al loro nonno; appartengono alla famiglia reale per via della loro nonna. Chiamarli, se avessero un cognome vero e proprio, con il cognome

Presidente, dovremmo chiederci il perché di questo disegno di legge

A prima vista può sembrare un disegno di legge che nasce da una risoluzione del Consiglio d'Europa, che affermava l'incompatibilità delle discriminazioni di genere nella scelta del nome di famiglia con il principio di uguaglianza di uguaglianza e raccomandava agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai propri figli.

è una profonda differenza tra una strutturazione che si riferisce ad un modello comunitario e una strutturazione che si riferisce ad un modello societario, cioè di società. Quello comunitario è un sistema di organizzazione coeso, che si fonda sulla solidarietà. Quello della società è un sistema di organizzazione che ha rapporti più labili,

quello organico e quello destrutturato. Quello destrutturato, in realtà, deriva da una visione del mondo che tende a recidere le radici (non a caso, poi, il cognome flessibile, in realtà, recide le radici), a destrutturare la famiglia e, soprattutto, a privare e a depotenziare le identità. Partiamo anche da una visione ampia: che cos'è la globalizzazione? La globalizzazione è una visione dei rapporti economici e sociali complessivi di una organizzazione sociale che è antagonista

tra vari modelli di Paesi ed ecco che, allora, il lavoratore italiano o francese dovrebbe essere competitivo come salario e livello produttivo con un lavoratore cinese o indiano. Questi modelli di prospettiva dello sviluppo delle comunità si stanno fronteggiando. quindi, che in un modello che si identifica con una società strutturata ci sono legami interumani che sono duraturi. È chiaro, invece, che in altri modelli i legami interumani diventano fragili e temporanei, cioè flessibili. è, allora, il modello di società che si va delineando per noi, in Occidente? È l'incubo della società liquida, l'incubo di una società nella quale tutto è flessibile. Una società nella quale la vita individuale diventa un progetto a breve termine. È una società nella quale si passa dalla conformità alle regole alla flessibilità. È chiaro che in questo tipo di società,

In altri modelli di società, che si rifacevano a modelli di vita che avevano progetti non a breve termine,

siamo rassegnati a prendere per buona e accettare qualsiasi idiozia ci viene proposta da Bruxelles.

A Bruxelles, dove si è rinnegata l'identità giudaico-cristiana dell'Europa, si è detto che bisognava realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome perché si parte dalla vecchia concezione della donna subalterna all'uomo. Vediamo se è davvero così.

A Sparta il lavoro delle donne non era certamente inferiore a quello degli uomini. La tradizione epica della Grecia e della sua cultura, mi riferisco all'*epos* omerico, parla di parità di rapporto tra i sessi, non di discriminazione. Per quanto riguarda la stessa costituzione di Licurgo, rifacendoci ancora non c'era questa discriminazione perché le donne potevano partecipare anche ai processi decisionali della città. Non a caso, nel 400 a.C. alle donne era possibile partecipare ai giochi olimpici. Quindi, non solo le donne partecipavano alle scelte importanti della comunità,

Quindi, quando in Occidente affermiamo che la nostra civiltà nasce dalla discriminazione della donna, da un ruolo subalterno di questa da una negata eguaglianza tra uomo e donna noi non consideriamo quali sono le radici della nostra civiltà.

su questo disegno di legge? Esso, dopotutto, trae origine da una frettolosa lettura del diritto comparato in ordine ai rapporti familiari in Europa. Certo, in Spagna esisteva la tradizione del cognome paterno seguito da quello materno: ma era, appunto, la tradizione di quel popolo;

d'Europa. Ma anche in Italia, con la normativa vigente, è possibile acquisire il cognome della madre affianco a quello del padre, in quanto si tratta di una libera

Ma, appunto, è una libera scelta. Quindi, noi potremmo optare per un indirizzo normativo che punti a liberare e a rendere molto più leggera sul piano burocratico la scelta relativa all'opzione di affiancare al cognome del padre anche quello della madre.

si arriva alla conciliazione corporativa dei due cognomi. Con questo, sostanzialmente, si torna ad un approccio

un approccio conflittuale tra marito e moglie nell'attribuzione del cognome? Dobbiamo ora soffermarci anche sull'approccio complessivo di un'area politica e culturale, la quale individua il conflitto sempre e dovunque.

mentre noi sappiamo che nella tradizione giudaico-cristiana l'uomo è custode della natura e non la aggredisce. Poi c'è il conflitto classico, marxiano,

nell'attribuzione e nella scelta del cognome, con la possibile priorità di un cognome su un altro. Si tratta di un altro elemento tipico della cultura della disgregazione. Signor Presidente, qui non si tratta di soffermarci a discutere di un disegno di legge

alle persone di attribuirsi un cognome, di rientrare in questo tipo di flessibilità familiare: qui si tratta di opzioni, di modelli di società.

Questo è un disegno di legge che propone il modello futuro della società destrutturata. Altri, come noi, propongono invece un modello un modello di società che non è quello tradizionale, ma affonda le sue radici nella cultura complessiva antropologica dell'Occidente. Qui noi non vogliamo confrontarci con le culture dei popoli. Il collettivismo, al limite, era proponibile come modello di sviluppo della società

sul villaggio contadino in cui esisteva la proprietà collettiva dei beni di produzione. Quindi, il collettivismo era già insito in quella società. Lo stesso totalitarismo marxista‑leninista cinese si modellava su un tipo di società che vedeva il mandarinato nascere da una burocrazia imperiale che si fondava sulla capacità di conoscere la scrittura e di praticarla, cioè sono modelli di società che hanno precise identità e in cui anche l'ipotesi marxiana trovava comunque una sua affinità, ma poi nel comunismo

di società che una parte maggioritaria di questo Paese respinge, perché la questione del cognome flessibile è identica a quella della famiglia flessibile dei DICO. Allora, se si ha questo modello di società liquida, che poi è un incubo perché è una società nella quale i legami interumani duraturi non esistono più, si scelgono i cognomi flessibili e la famiglia flessibile, se ci si riferisce ad un altro modello di società si

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se c'era un provvedimento per tenere impegnato il Senato nel segno dell'Unione è quello che stiamo discutendo - non a caso è stato presentato da esponenti dell'Ulivo e di Rifondazione

parte dell'Unione Europea, l'emergenza rifiuti in Campania ben più drammatica, oppure sulla vicenda parlamentare ancora più rilevante Visco-Guardia di finanza - guarda caso - su cui occorrerebbe fare chiarezza al più presto. Se c'è un problema di cui gli italiani e di cui il Paese non hanno bisogno è questo disegno di legge in materia di cognomi. Il cognome è quella parte del nome di una persona che indica a quale famiglia appartiene. L'uso del cognome si fa risalire all'antica Roma: dopo la caduta dell'Impero romano, ogni persona veniva identificata sulla base del suo nome personale; con la grande crescita demografica tra il X e l'XI secolo divenne complicato distinguere un individuo col solo nome personale e si pose il problema

per distinguere le sepolture, i matrimoni, i battesimi, e anche l'obbligo per i parroci di gestire un registro con nome e cognome al fine di evitare matrimoni tra consanguinei per gli effetti che ne potevano derivare?

che vanno dai DICO all'eutanasia camuffata da testamento biologico, al cambiamento appunto del cognome e che rappresentano un attacco concentrico alla famiglia. E pensare che questa maggioranza aveva creato un Ministero a tutela della famiglia, quale contraddizione più evidente! Ma di quale famiglia si vuole parlare? Invece di dare risposte concrete alle famiglie che hanno fatto sentire la loro voce con il *Family day*, quella straordinaria manifestazione di popolo e di testimonianza dei movimenti laicali-cattolici nella modernità, invece di preoccuparvi della pesante pressione fiscale per le famiglie, di abolire o quantomeno ridurre l'ICI per la prima casa, di dare di dare competitività alle imprese, di offrire servizi che funzionino, di assicurare la puntualità dei treni e degli aerei e di ogni mezzo di trasporto, di determinare efficienza e semplificazione nella pubblica amministrazione, ponete questa questione come prioritaria e centrale per lo sviluppo del Paese. La vostra scelta va, invece, nel senso di distruggere l'istituto familiare in nome di un individualismo imperante ed esasperato. Tutto ciò è un retaggio post-sessantottino che volete affermare in nome di una presunta modernità, di una presunta e falsa idea di progresso, che abbatte le formazioni intermedie e realizza il principio di uguaglianza per altri fini subdoli, intervenendo su una materia complessa come è l'attribuzione del cognome ai figli. Del resto, è stato ribadito in Commissione che privilegiare il cognome materno significa tradurre sul piano normativo una tendenza culturale tesa a valorizzare il ruolo della donna nella storia familiare. Questo concetto lo abbiamo sentito riecheggiare anche nel corso del dibattito e se prevale il «fai da te» dove finisce l'unità del nucleo? Non è questione irrilevante per i bambini portare il cognome dei genitori anche per collocarli nel sistema delle parentele. Voi, invece, volete l'esaltazione dell'individualismo anziché del gruppo parentale, ed allora è bene essere chiari: dopo 2.000 anni di diritto romano volete scardinare un istituto millenario per inseguire culture estranee alla nostra tradizione, aggiungendo tensioni che già si manifestano, per esempio, quando si tratta di scegliere il solo nome del neonato, se si vuole rispettare la tradizione di ricordare la figura del nonno o della nonna. Fate prevalere l'ordine alfabetico come criterio di scelta in caso di controversia. E perché non prevedete il ricorso al sorteggio, come nell'antica Grecia, con metodo autenticamente democratico! Poiché siete contro la famiglia intanto cominciate a distruggerla con il cognome. Forse a voi basta solo un numero come quello delle agenzie fiscali. È allora una questione culturale prima ancora che politica. Volete annullare Storia e radici, anticipando i DICO con l'assemblaggio dei singoli. Combattete a parole la precarietà del lavoro e poi la esaltate con le unioni parafamiliari e nella trasmissione dei cognomi, come con la previsione di dichiarazione congiunta all'atto del matrimonio e poi prevedendo precarietà nelle vicende della vita familiare, mutate le scelte originarie con dichiarazioni revocabili. Guarda caso, strana similitudine con i DICO! Anche lì bastava una raccomandata! L'Unione fa scomparire la famiglia e fa nascere l'unione di individui. C'è anche un aspetto costituzionale che va rilevato: quello delle formazioni intermedie, costituite dai Comuni, dalle famiglie, dalle comunità territoriali e familiari, promosse dai costituenti. Al riguardo va citato l'ordine del giorno Dossetti,

tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome, singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto all'articolo 22 della Costituzione, che assume la caratteristica del del segno distintivo e identificativo della persona nella sua vita di relazione accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, e costituisce parte essenziale e irrinunciabile della personalità. Dimenticate il problema dei figli, che per noi sono figli della famiglia, mentre secondo voi sono del singolo o di un solo genitore, distruggendo l'unità del nucleo. Il ministro Bindi dovrebbe dedicarsi a risolvere i problemi delle famiglie, non solo con manifestazioni propagandistiche, ma con interventi seri, e questa è una questione seria. Il cognome è identificativo della famiglia e della discendenza e voi volete risolvere un problema così complesso con questo curioso "mostriciattolo", come lo ha definito acutamente il senatore Massimo Livi Bacci. I genitori avrebbero quattro possibilità: imporre al figlio il cognome del padre, quello della madre o ambedue in ordine padre-madre o madre-padre. Alla terza generazione i poveri fanciulli avranno la bellezza di 32 cognomi, cioè - appunto - una moltiplicazione dei cognomi. II percorso generazionale diventerebbe una gincana onomastica, della quale non si capiscono né il significato né l'utilità, mentre la storia del cognome come identificativo di una famiglia e di una discendenza è di grandissimo interesse sociale. Sarebbe bene far prevalere un minimo di saggezza rispetto a questo pasticcio genetico che alimenta solo confusione.

II Parlamento sta predisponendo distrattamente, potremmo dire nel silenzio più assoluto, la modifica di articoli importanti del codice civile relativi al cognome della moglie e dei figli. Si tratta di una rivoluzione di princìpi che hanno una millenaria tradizione, che va al di là dei profili strettamente anagrafici, sconvolgendo - appunto - princìpi secolari. L'unica questione aperta sembra essere l'ordine precostituito o casuale con cui dovranno apparire entrambi i cognomi dei genitori: questo argomento sembra appassionare molti, ma non certamente coloro che hanno a cuore i veri problemi della famiglia. Desta non poche preoccupazioni il tentativo di innovare radicalmente una tradizione, senza che la problematica relativa sia stata adeguatamente dibattuta e senza neppure che la disciplina in vigore costituisca deroga al principio di parità morale e giuridica fra i coniugi posto dall'articolo 29 della Costituzione, atteso che lo stesso articolo consente limitazioni funzionali all'esigenza di garantire l'unità familiare. È poi così urgente questo tipo di intervento? Non sarebbe più urgente e proficuo che il Parlamento desse priorità ai temi della condizione economica di una larga parte delle famiglie italiane, della devianza minorile, delle provvidenze anche economiche necessarie perché vengano adempiuti i compiti che ai genitori assegna l'articolo 30, comma 1, e che sono ribaditi dall'articolo 31 della stessa Costituzione? Onorevole Presidente, si dovrebbe cercare di recuperare un minimo di sobrietà, di serietà e soprattutto di prudenza e si dovrebbero evitare demagogie.

definisce l'attribuzione del cognome del padre un retaggio della concezione patriarcale della famiglia. La definizione "patriarcale" della Corte ovviamente si riferisce alla famiglia come istituto giuridico del nostro ordinamento, proprio a quella società naturale che è stata, in questo stata, in questo momento politico e culturale, da parte di molti esaltata e richiamata proprio per la sua naturalità. Viceversa, l'aggettivo patriarcale dovrebbe obbligarci tutte e tutti a prendere atto del carattere storico, sia pure nei mutamenti e nell'evoluzione, della storia di una civiltà, dell'istituto famigliare. Direi di più: il termine patriarcale nomina l'origine stessa della famiglia, a cosa si deve proprio il costituirsi di quel nucleo che ne ha rappresentato la continuità nel corso di secoli e di millenni, continuità che trova il suo suggello, il *signum* simbolico e sociale, proprio nel cognome materno, (*lapsus* significativo). Infatti, la famiglia patriarcale - è bene insistere su questo aggettivo non solo è storica, come tutti gli istituti giuridici, è una costruzione artificiale dovuta alle leggi e ai costumi umani, ma nella sua origine, tra tutte le istituzioni umane, la famiglia nasce nasce contro natura, è un istituto contro natura, come tale è stata tramandata e come tale ha avuto un posto centrale nelle società e nella civiltà. Contro natura, infatti, sono i rapporti di parentela, in particolare quelli di discendenza, le genealogie sociali e simboliche che si pretenderebbe che si pretenderebbe e si presume - e su questo si è costruita un'intera cultura - corrispondano ai rapporti naturali, ma in realtà si fondano proprio sul loro rovesciamento, sulla negazione del nucleo di naturalità che c'è nella relazione tra i sessi, tra l'uomo e la donna nella procreazione e nella relazione tra genitori e figli. La famiglia nasce, infatti, per dare una risposta, con la legge degli uomini, a quella che appariva una delle poche evidenze dell'esperienza umana agli albori della società, questa sì naturale: quella che si nasce da donna e che la relazione con la madre è la vera relazione primaria, che inizia ancor prima della nascita. Le leggi degli uomini, le leggi sulla famiglia, ma anche le leggi sulla che hanno costituito la città politica, gli Stati, hanno affermato il diritto e il potere del padre come diritto dell'uomo sui figli e come diritto e potere dell'uomo sulla donna: questa è stata la patria potestà, che è stata cancellata ieri, rispetto a questi tempi storici, nel 1975, e questo diritto-potere del padre è ancora espresso proprio nel cognome. Ancora oggi esistono istituti nel nostro ordinamento - ne cito uno tra tutti: la paternità presunta - che affermano la supremazia della posizione del padre rispetto alla madre. Penso che il cognome sia stato storicamente il principale strumento politico, vorrei dire strategico, con cui gli uomini hanno regolato la sessualità e la procreazione, hanno costruito attorno alla famiglia alleanze sociali ed economiche, hanno esercitato il controllo sul corpo delle donne ed hanno esercitato la potestà sulle donne e sui figli, hanno governato la trasmissione di patrimoni, di tradizioni culturali, di identità, hanno fatto la storia delle generazioni. È l'uomo a istituire il legame anche con la madre, proprio perché - come ancora è registrato nel codice e in questa legge si propone comunque di segnare un mutamento, un passo avanti - esiste la distinzione tra figli legittimi nati nel matrimonio e figli che ieri si chiamavano illegittimi, oggi naturali, e che il disegno di legge propone di definire nati nel e fuori dal matrimonio, ma comunque la distinzione permane. È l'uomo che ha assegnato proprio con il cognome il posto di chi nasce nelle relazioni sociali. La sentenza della Corte costituzionale indica una via per rimuovere questo retaggio patriarcale del cognome nel principio dell'uguaglianza tra donna e uomo. La soluzione che come tale si prospetta prospetta come la più rispondente a questo principio è quella del doppio cognome, come regola bilanciata con la libertà dei genitori di decidere l'ordine dei cognomi e quale trasmettere. Ma c'è da fare una osservazione anche rispetto a questa soluzione, ad assumere cioè l'uguaglianza come il principio che ci permetterebbe davvero di fare giustizia di questa storia del patriarcato e di portare ad una maggiore corrispondenza le relazioni naturali e quel nucleo che c'è nella sessualità e nella procreazione di naturalità con le norme giuridiche. Non dobbiamo infatti mai dimenticare, e invece continuamente viene negato, che non c'è parità tra uomo e donna nella anzi il contrario. La scelta di un uomo di avere un figlio dipende oggi come ieri dalla volontà di una donna di divenire madre. Dico oggi come ieri perché, in un contesto segnato dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita, non vi è ancora modo - nessuna tecnica lo può fare perché ad un concepimento segua davvero la nascita di un figlio. E da sempre, proprio da sempre, nonostante i divieti, le leggi e i controlli che gli uomini hanno posto sul corpo delle donne, non vi è modo - non vi sarà modo di imporre ad una donna per legge se e come divenire madre. Il Gruppo di Rifondazione Comunista ha sostenuto, nel dibattito in Commissione, Commissione, la proposta di legge presentata dal presidente Caprili, quella che molto semplicemente fa giustizia, rispetto alla storia dei rapporti, proponendo che chi nasce assuma il cognome della madre. madre. Diversamente dalla sentenza della Corte costituzionale, se il principio dell'uguaglianza può essere ritenuto condivisibile per quanto attiene alla condivisione da parte della della madre e del padre dei diritti e doveri nei confronti dei figli, questo principio andrebbe bilanciato - cito dalla relazione del presidente Caprili al suo disegno di legge - con il riconoscimento dell'inalienabile priorità della relazione della madre con i figli e con le figlie. Questa sarebbe la sola scelta che davvero rispetta l'ordine delle relazioni naturali, la sola che potrebbe fare giustizia rispetto alla storia millenaria del patriarcato. Ma sono consapevole - credo che tutti i senatori e le senatrici del mio Gruppo lo sono - che questa scelta, proprio per la radicalità e per l'andare alla radice (nel senso etimologico) del problema, incontra resistenze sedimentate in una lunga tradizione. Penso che possa essere una soluzione condivisibile ed accettabile quella del doppio cognome se alla scelta del doppio cognome la formulazione che viene adottata

prospettare una soluzione, favorire la sua adozione nei comportamenti sociali. Quindi, ci deve essere una regola nel doppio cognome, una regola però bilanciata che faccia salva la scelta della madre e del padre di poter definire l'ordine dei cognomi, di preferire quello della madre, della donna, a quello del padre. In questa direzione pensiamo che adottare una legge, diversamente da quello che è stato detto in molti interventi, corrisponda ad una richiesta diffusa nella società, anche se non si esprime come una urgenza perché - vorrei ricordare - uno dei mutamenti più profondi che le nostre società conoscono è proprio quello dei rapporti tra uomini e donne. La rivoluzione femminile è una di quelle che sta segnando un'epoca. Se noi non vogliamo che tale rivoluzione veda il nostro ordinamento arroccato nella conservazione e addirittura destinato per questo ad arretrare, dobbiamo

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si affronta il problema onomastico, si affronta il problema dell'identità della persona. Trattandosi di cognome, noi dobbiamo scegliere dunque tra una identità chiara, forte, non transitoria, ovvero un'identità debole e continuamente mutante. È il problema, d'altro canto, più generale, degli uomini e delle donne di oggi sapere chi siamo e da dove veniamo o non avere un passato, avendo dunque un presente confuso e un futuro incerto e problematico. Una identità soggettiva forte presuppone una famiglia forte, unita, stabile, a cominciare dalla consapevolezza della sua storia e della sua identità. Una volta la famiglia era il primo luogo di trasmissione di valori che si tramandavano di generazione in generazione. Oggi ciò avviene con sempre maggiore difficoltà, ed è anche per questo che la nostra società è in crisi. La proposta di legge che qui discutiamo distrugge l'identità familiare, non fornisce infatti alcun criterio legale e delinea una soluzione, quella dell'ordine alfabetico, che potrebbe portare a soluzioni aberranti, come quella di un tale che si chiama Verdi, suo figlio Rossi e il nipote Bianchi. La scelta del cognome è fatta discendere da una mera casualità. A prescindere dai dubbi di costituzionalità di una scelta certamente irragionevolmente discriminatoria, il suo obiettivo è quello di rendere ancora più flebile l'identità familiare. Il carattere transitorio della famiglia dipende anche dalla possibilità, per il figlio, di rimettere continuamente in discussione, senza motivi significativi e forti, la scelta fatta dai genitori. Ma la soluzione Ma la soluzione di non fornire alcun criterio legale e di rimettere tutto alla decisione degli sposi introduce anche un elemento di potenziale conflittualità che rischia di far entrare in crisi il matrimonio fin dal suo sorgere. Ancora più grave è il fatto che la scelta, fatta nell'atto di matrimonio, possa essere revocata e sia possibile modificarla ancora nell'atto di nascita. Qui si offrono armi a ricatti continui, ad una occasione di scontro procrastinata nel tempo. D'altro canto è giusto rispettare, com'è stato da più parti sottolineato, la nostra millenaria tradizione ma è altrettanto giusto, anzi è doveroso, garantire anche alla donna la possibilità di trasmettere al figlio il proprio nome. Sarebbe a mio avviso rozzo ed ottuso maschilismo negare alla donna la possibilità di dare al proprio figlio anche il proprio cognome. Un conto è disgregare l'identità della famiglia senza fornire un criterio legale automatico, un altro è considerare la donna come un soggetto non titolare di un diritto alla trasmissione onomastica, come se fosse un soggetto giuridicamente inferiore, E comunque, che piaccia o no, vi è una sentenza della Corte costituzionale e dunque una risposta va data. Io ho fatto una proposta di emendamento su cui ho registrato una convergenza molto ampia: fornisce un criterio legale, un criterio che rispetta

Dato che si tratta di una materia molto delicata, si approfondisca pure questa soluzione, purché non la si peggiori, né la si complichi. Personalmente auspico comunque una scelta che parta da un criterio legale certo e non eversivo, che garantisca la continuità della famiglia e che, nel contempo rispetti il diritto della donna di dare anche lei al proprio figlio il proprio cognome. Questa è una soluzione equilibrata, non è ideologica, e credo soprattutto che sia una soluzione di buonsenso.

Signor Presidente, siamo qui dopo circa due mesi di cassa integrazione, un istituto nuovo per quanto riguarda il Parlamento, cassa integrazione nella quale il Governo e la maggioranza ci hanno costretto.

all'attività politica e al rapporto con i cittadini. In questi due mesi di cassa integrazione si è alimentata una polemica nei confronti della politica, del Governo, delle istituzioni, ma più in generale di tutta l'attività politica e della rappresentanza che ha coinvolto ed in qualche misura travolto dai mezzi di comunicazione di massa

quella sì, ben nutrita di privilegi di corporazione. Alcuni di loro - quelli che si occupano della casta dei politici - sono una casta nella casta: infatti, perché i giornalisti del «Corriere della Sera», Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella in particolare, godono forse di privilegi più duraturi e più solidi di quelli che loro attribuiscono a chi fa politica o ai parlamentari. In questi due mesi di sospensione la difficoltà a controbattere a tali argomentazioni era enorme. E ancora più enorme si è fatta adesso, dopo i due mesi di cassa integrazione, quando numerosi mi hanno chiamato e mi hanno detto: bene, adesso ci sono state le elezioni. C'è un terremoto politico. Il Paese richiede una serie di provvedimenti e di cambiamenti urgenti.

di cognomi: se questa è la risposta che le istituzioni ed il Parlamento danno ad un momento di difficoltà obiettiva della Nazione, ebbene si alimenta il discredito e la scarsa considerazione che nel Paese si ha delle istituzioni stesse. Credo quindi, Presidente, che se è vero quello che ha detto ieri il presidente Marini, che questo provvedimento ha comunque una sua dignità, questo vale ovviamente per tutti i provvedimenti. Però non credo che la nostra missione, il nostro privilegio di rappresentare il popolo sia ben esercitato dilettandosi in queste modifiche al codice civile, che mi pare nessuno attendesse come panacea di qualche male. Dopo questa premessa di metodo, voglio entrare nel merito dei provvedimenti.

di problemi che anche le manifestazioni popolari hanno sollevato rispetto alla condizione materiale e al riconoscimento delle funzioni sociali della famiglia, occuparci dell'onomastica mi sembra non il migliore dei punti di partenza. Ma voglio entrare ancora più nel merito di questo provvedimento. Se noi lo esaminiamo nelle sue singole norme, in fondo non ci sarebbe quasi nulla da obiettare.

Non lo so, sarà per ragioni corporative, ma io sono sempre un po' in fondo negli ordini alfabetici e quindi rischierei in questa situazione di veder disperso il mio cognome in base a qualcosa su cui potremmo intervenire la prossima settimana.

È la filosofia per la quale, per esempio, un soggetto che soffre di un'inabilità per un problema fisico viene chiamato portatore di *handicap*, non handicappato, trasferendo su di lui l'inabilità come difetto e non riferendosi al fatto che se incontra un ostacolo ne viene handicappato. viene handicappato. Oggi sono arrivato all'ultimo minuto perché sono stato handicappato a trovare il parcheggio per la mia auto dalla presenza di numerose scorte di membri del Governo: questo è un *handicap* esterno. Una persona che ha un problema di deambulazione ha il problema di superare ostacoli troppo grandi: un *handicap* esterno. No, la filosofia del *politically correct*, siccome handicappato suona male, lo chiama portatore di *handicap* e così gli rovescia addosso il problema che prima invece apparteneva alla società. In questa ideologia *politically* *correct* del nome delle cose,

di scegliere il nome del padre o della madre il significato dell'uguaglianza nell'ambito della famiglia. Ma lei crede, Presidente, che se i figli di quell'uomo che è stato arrestato ieri a Perugia non si fossero chiamati Spaccino ci sarebbe stata una condizione di uguaglianza in quella famiglia, in quella famiglia, perché magari i figli avevano preso il cognome di quella donna uccisa? O forse nelle famiglie esistono problemi che vanno molto più in profondità, sono molto più seri e per risolvere i quali questo Parlamento dovrebbe in qualche modo agire, piuttosto che occuparsi, e così approfonditamente, di un tema solo perché questo è frutto di una convenzione internazionale, che a sua volta ha avuto ricadute in altri Paesi, che hanno risolto il problema in diversi modi, fino a che noi non abbiamo trovato le agili soluzioni proposte in questo disegno di legge? La mia opposizione, la mia contrarietà a questo disegno di legge è rivolta tutta alla filosofia del *politically* *correct.* a volte ho l'impressione, quando entro in quest'Aula dopo essere stato due mesi nel mondo reale (che mi hanno aiutato), di essere su *Second life*. Non so se lei ha presente quel mondo virtuale a cui si accede da Internet, nel quale ciascuno di noi può attribuirsi l'identità che vuole e costruirsi intorno il mondo che vorrebbe, facendolo interagire con i mondi che altri vorrebbero. *Second life* è un bellissimo gioco ed è un *divertissement* virtuale che sta coinvolgendo milioni di persone. Non capisco, però, perché le istituzioni debbano essere una *Second life*. Noi qui ci stiamo occupando del *second surname* - mi permetta il gioco di parole, visto che siamo su *Second life* - e non ci stiamo occupando, invece, di ciò di cui ci dovremmo occupare. Dovremmo occuparci, per esempio, del fatto

nei consensi. Da che cosa è dipeso? L'hanno detto chiaramente: è colpa del Governo, la responsabilità è tutta del Governo. Ebbene, forse dovremmo discutere del fatto che il Governo si manifesta inadeguato

non vedono riconosciuta la propria funzione sociale e sono spesso il centro dell'assistenza a cui le costringiamo, a causa della distorsione del nostro sistema economico, per il quale

quali sarebbero dovuti entrare per portare lavoro e invece ricevono benefici e assistenza. Alle famiglie che cosa diamo, di fronte a queste difficoltà

provoca, però, un'ulteriore ondata di discredito sulle istituzioni, sulla politica, di fronte ad un Paese che è in difficoltà, che reclama a gran voce un mutamento nell'indirizzo politico, che viene spesso aizzato ad additare come responsabili tutti, in modo indistinto, come se non esistessero

Il popolo ha dato prova di come vuole mutare l'indirizzo politico. Ebbene, signor Presidente, occorre urgentemente mutare l'indirizzo politico del Paese, cambiare l'attuale situazione; occorre che il Governo

il relatore, senatore Salvi, ha fatto riserva di ulteriori messe a punto del provvedimento, anche con un eventuale ritorno in Commissione, sulla stregua delle risultanze del dibattito svolto in Aula fra ieri sera e stamani. Perciò, intervengo ora, in sede di discussione generale, soltanto per anticipare un'intenzione di voto che deriva totalmente dalla questione di principio. Le poche cose che dirò riguardano la scelta di principio, salvo le ulteriori considerazioni che si potranno fare, quando sarà il momento giusto, nel merito specifico delle norme. Dal dibattito che abbiamo ascoltato sono emerse una serie di obiezioni che, per la verità, non mi sembrano tutte di portata decisiva. Con tutto il rispetto per il senatore Eufemi, non vedo come provvedimenti quali i diritti dei conviventi, la dichiarazione anticipata di rifiuto dell'accanimento terapeutico e i cognomi dei figli possano costituire un trittico, trattandosi di tre provvedimenti totalmente disparati nel loro contenuto e nella loro intenzione. Così ancora non mi sembra decisiva l'obiezione - ritornata peraltro in una pluralità di interventi - circa il fatto, di per sé innegabile, che anche in materia di sostegno alla famiglia vi sono emergenze legislative più pressanti di quella di cui ora si discute. Ciò è stato sostenuto da molti senatori dell'opposizione,

è altrettanto fuori di dubbio che al Senato, se vuole, non manca il tempo per occuparsene. Penso, invece, che nella stentata produzione normativa del primo anno della XV legislatura poche leggi, come quella che oggi si discute, rientrino a buon diritto nella categoria delle leggi di riforma. E si tratta molto significativa, nel senso che modifica una tradizione giuridica ed un costume sociale secolari, per qualche aspetto millenari: la tradizione e il costume di chiamare i figli con il cognome del padre. Voglio raccogliere un'osservazione che ho ascoltato stamani dal senatore Malan, circa il diritto derivante dalla consuetudine. Quanto quella tradizione e quel costume di attribuire ai figli il cognome del padre siano radicati è provato dal fatto che la consuetudine non richiede neppure una norma esplicita e il fatto di riformare un uso, che affonda le radici nel diritto romano, chiama in causa una prima questione di principio piuttosto importante nella filosofia del diritto di impronta liberale. Mi riferisco alla teoria liberale del diritto e della legge che si riconduce, tra gli altri, a Friedrich Von Hayek, un autore il cui pensiero presumo il senatore Salvi non condivida molto, ma che ma che sicuramente conosce, e che, d'altra parte, ha avuto anche corrispondenze significative nella filosofia del diritto italiana, segnatamente e anche in forme più radicali di quella seguita da Hayek, nel pensiero di Bruno Leoni. Tale teoria considera il diritto, in analogia un poco con il linguaggio, come un processo di sedimentazione, che si forma per consuetudine condivisa e che la volizione del legislatore dovrebbe modificare solo con rallentata prudenza. L'uso di trasmettere ai figli il cognome del padre appartiene, come molti giustamente hanno detto, alla potestà antica del *pater* *familias*. Nella Roma classica mi sembra che anche i senatori si chiamavano *patres*. La riforma porterà, modificandola, anche a qualche complicazione pratica. è prevedibile che nell'arco di qualche generazione le scienza della genealogia e dell'onomastica diventeranno scienze difficili.

è già molto cambiato rispetto alla normativa codicistica che, a presidio della potestà maritale, obbligava la donna a seguire il marito subendone anzitutto il cognome. Da più di trent'anni la riforma del diritto di famiglia mantiene alla donna il cognome di nascita, solo aggiungendovi il cognome del marito. Il fisco, per la verità, non applica neppure questa Tuttavia, anche in quel modo, il cognome del marito resta l'unico in comune alla famiglia fondata sul matrimonio e, in quanto tale, l'unico a trasmettersi ai figli. il principio che adesso entra in gioco è di stabilire, anche nel nome, la parità fra i coniugi e, ciò che più conta, dei coniugi nei confronti dei figli. la riforma intende stabilire anche nel nome, diritto protetto dalla Costituzione, la parità dei generi, essa deve rimuovere l'ultimo residuo della potestà maritale, seguendo l'indirizzo indicato dalla Corte costituzionale. In che modo? Signor Presidente, non conosco la sua personale opinione in proposito, ma ho trovato apprezzabile la proposta di legge del senatore Caprili di rovesciare la trasmissione del cognome da quello paterno a quello materno in considerazione del dato di fatto che, nella generalità delle famiglie, è la madre la figura principale ed essenziale del vincolo di dedizione, di coesione e di unità, però questo darebbe luogo ad una disparità ribaltata e non alla parità. Per la stessa ragione, anche il testo sostitutivo dell'articolo 2, proposto dal senatore Livi Bacci, conserva tra i coniugi (salvo loro diverso ed eventuale avviso) una clausola prioritaria a favore del padre e, quindi, una disparità residuale. Invece, il senso riformatore della legge risiede interamente nella piena parità dei coniugi. Per tale motivo, condivido la proposta del relatore e considero la legge un atto di grande portata simbolica nell'attuazione del principio costituzionale di eguaglianza tra i generi. Salvo l'apprezzamento di ulteriori emendamenti che potranno essere portati al testo, in linea di principio anticipo il voto favorevole, con qualche rammarico per il fatto che la parità del cognome possa applicarsi soltanto ai primogeniti che nasceranno dopo la promulgazione della legge.

Vorrei fare solo due brevi considerazioni di ordine generale su alcuni temi che sono stati sollevati. Il primo concerne il riferimento all'articolo 29 della Costituzione.

C'era un'opinione la quale riteneva che la formula della società naturale dovesse rimandare all'immutabile - così veniva considerato - modello tradizionale della famiglia patriarcale, basata sul ruolo prevalente del padre, padre, sulla discriminazione tra figli legittimi e figli nati fuori del matrimonio (l'espressione che allora si usava era «figli illegittimi») e sulla prevalenza dell'uomo sulla donna. Ora questa tesi è stata superata da due fattori: l'introduzione della legge sul divorzio, che ha eliminato un elemento della tradizione plurisecolare della famiglia introduzione ritenuta legittima da una sentenza della Corte costituzionale - e in secondo luogo la riforma del 1975 del diritto di famiglia, che ha profondamente modificato il modello patriarcale di famiglia, valorizzando quelle altre norme costituzionali che, ispirandosi al principio di eguaglianza, fanno riferimento sia al rapporto tra l'uomo e la donna, sia alla pari tutela dei figli, siano essi nati nel matrimonio o fuori del matrimonio. riproporre una tesi per la quale invece l'articolo 29 della Costituzione debba intendersi riferito ad un modello tradizionale di famiglia, che da oltre trent'anni in Italia non esiste più,

sotto il profilo del principio di parità tra uomo e donna, una modifica della disciplina del cognome familiare. Questo punto è stato chiarito in modo inequivocabile dalla sentenza della Corte costituzionale, la quale fa seguito ad un'ordinanza di remissione della Corte di cassazione dal primo pretore di passaggio). I supremi organi giurisdizionali in Italia, che sono la Corte di cassazione e la Corte costituzionale (che non credo siano affette da volontà eversive nei confronti dell'istituto familiare), invitano quindi il Parlamento a modificare questa normativa, del tutto evidente che se non lo faremo noi, fra non molto tempo lo farà la Corte costituzionale adottando, fra le diverse soluzioni possibili, quella che riterrà più adeguata. Per quanto riguarda la questione delle priorità, vale a dire se sia questo il primo tema di cui occuparsi, la considerazione può riguardare qualunque argomento, qualunque materia. Vorrei ricordare che un'iniziativa legislativa in questo senso, anche se non è andata in porto, fu assunta nella passata legislatura dalla maggioranza di centro-destra, rammentando che fin dall'inizio di questa legislatura sono stati presentati diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare di cui la Commissione giustizia ha iniziato l'esame nel settembre dello scorso anno, dedicando loro otto sedute e approfondendo il tema. tema. Come ho già detto ieri, integrando brevemente la relazione scritta, e sulla base di quanto emerso dall'esito del dibattito, credo sia utile approfondire i punti emersi, anche perché la normativa ha una sua tecnicità che richiede un coordinamento complessivo delle norme.

la revisione comporta una ristrutturazione dell'intero disegno di legge, come ricordava anche il senatore Manzione nel suo interessante intervento. La senatrice Alberti Casellati ha posto a sua volta un tema che ha un certo rilievo, sul quale ha presentato anche un emendamento

L'emendamento da lei presentato pone la questione e credo che anch'esso vada approfondito dal punto di vista tecnico‑giuridico; anche questo è un contribuito che il che il Parlamento - e, se la mia proposta verrà accolta, la Commissione - potrà approfondire e verificare nei suoi aspetti tecnico-giuridici. Per queste ragioni, signor Presidente, credo sia opportuno un rinvio del provvedimento in Commissione in modo che in un lasso di tempo ragionevole, per esempio quindici giorni, la Commissione possa verificare, sulla base degli emendamenti che sono stati presentati in Senato e della discussione che si è svolta, è svolta, la possibilità - che a mio avviso esiste - di trovare una soluzione condivisa che il Senato stesso possa trovare nel suo insieme evidentemente preferibile a quella che era stata varata della Commissione.

LEGGE Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile ( GNSS ) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004

onorevoli senatori, siamo chiamati ad interessarci del disegno di legge n. 1331, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e lo Stato di Israele,

(appunto «*Global Navigation Satellite System*», d'ora in poi GNSS).

europea (ESA), un sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, così pervenendo al programma Galileo, quale sistema globale autonomo europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite ad uso civile. La realizzazione dell'ora detto programma si articola attraverso tre fasi: la prima, la prima, 2002-2005, ha riguardato la verifica e la messa a punto delle componenti dell'architettura del sistema; la seconda fase, 2006-2007, prevede il lancio dei satelliti (il primo è stato posto nell'orbita il 28 dicembre 2005), nonché l'installazione delle strutture terrestri;

Circostanza di rilevante interesse sotto il profilo dell' economia dei costi, oltre che sotto l'aspetto delle semplificazioni tecniche e tecnologiche, è la compatibilità tecnica e l'interoperatività nel progetto Galileo con il sistema statunitense di radionavigazione via satellite «*Global Positioning System*» - GPS - gestito dalle autorità militari statunitensi. Galileo è un «Programma» aperto a collaborazioni internazionali con Paesi terzi. Esso è iscrivibile, quindi, nel quadro delle collaborazioni internazionali avviato dalla Comunità europea con Stati terzi. In questo contesto giova ricordare che l'Accordo con Israele, di cui ci stiamo occupando, segue quello con la Cina del 30 ottobre 2003, e quello con gli USA del 26 giugno 2004, ed è stato seguito da quello con l'Ucraina, il 3 giugno 2005. giova menzionare che sono stati inoltre parafati analoghi accordi con l'India e il Marocco, rispettivamente nel settembre e novembre 2005. Come per gli altri Paesi che aderiscono al progetto Galileo, anche per quello di cui ci stiamo oggi occupando è prospettabile una significativa opportunità sotto il profilo della collaborazione tra TUE ed Israele in più settori scientifici e tecnologici, dell'ambiente e dell'energia, dell' industria, dell'agricoltura e della pesca, dei servizi, della medicina.

dell'attenzione sul tema da parte dell'Aula, per quanto riguarda il merito delle convenzioni - ripeto - già sottoscritte dall'Unione Europea con Stati terzi, lo schema dell'Accordo ripete schemi precedentemente già esaminati. Pertanto, nel merito

che, inerentemente all'accordo, hanno espresso parere essenzialmente favorevole le seguenti Commissioni: 1a,4a, 7a , 10a

conferendomi all'unanimità mandato a riferire in tal senso all'Assemblea. Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di tre articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sopra esaminato, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge. Si propone l'approvazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione

con gli Stati Uniti d'America. Galileo è il programma europeo più importante di radionavigazione e di posizionamento via satellite. Si tratta di una tecnologia, tutta europea, di punta. Galileo rappresenta il primo grande progetto industriale spaziale dell'Unione Europea; si inserisce pienamente nella Strategia di Lisbona ed è, quindi, il primo Sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare disegnato per uso civile a livello mondiale. L'accordo con Israele fa parte dell'iniziativa volta ad estendere a Stati terzi questo progetto e questa tecnologia. Simili accordi sono stati siglati con la Cina, gli Stati Uniti, l'Ucraina, il Marocco, l'India e la Russia. L'Unione Europea ed Israele intendono collaborare sia bilateralmente che nelle sedi multilaterali per promuovere e facilitare l'uso del sistema di navigazione GPS. Credo che, tra l'altro, ciò si inserisca nell'attività più generale di cooperazione, nella cornice dell'Accordo Euro-Mediterraneo Unione Europea ed Israele, che è il nostro principale riferimento.

Signor Presidente, anch'io mi congratulo con il relatore per l'attenzione, per la specificità e per la precisione con cui ha illustrato

tra i Paesi civili e democratici del mondo è isolato quanto lo Stato di Israele. Tale Paese non fa parte di alcun gruppo o di alcuna aggregazione nell'ambito delle Nazioni Unite e - al di fuori del particolare rapporto

degno di nota perché è unico, se pensiamo ad un'infinità di situazioni discutibili nel mondo. Si pensi a Myanmar, l'ex Birmania, che tiene in prigione da venti anni la vincitrice, premio Nobel, delle elezioni democratiche di quel Paese, e fa parte di tutte le aggregazioni e i gruppi possibili alle Nazioni Unite; oppure, si pensi al Sudan del Darfur e così via. Sarebbe un lungo elenco. Israele è isolato e questo è un trattato che ci dà l'occasione di diminuire quell'isolamento e quella solitudine. È dunque una ragione in più, oltre a quelle che ha portato con perizia e con precisione il relatore, oltre alle dichiarazioni che ha appena reso il Governo, per dire sì

mi dilungherò troppo, ma credo che sia importante - benché il collega Bianco ed io abbiamo già presentato la relazione scritta che che potrete consultare - porre il provvedimento in un quadro più generale. Il testo è stato esaminato dalle Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro e previdenza sociale, e debbo dire che questo disegno di legge, nel testo che qui è sottoposto alla vostra attenzione, ha ricevuto una larga approvazione in sede di Commissione, con una confluenza di opinioni molto larga della maggioranza e dell'opposizione, quindi ringrazio del lavoro collaborativo che è stato svolto in Commissione. Vorrei dare, molto brevemente, un quadro generale e ricordare che questo provvedimento riguarda interventi per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori che sono irregolarmente presenti nel territorio e che il nostro Paese ha un grado di irregolarità la sanatoria del 2002-2003 ha sanato le posizioni di più di 600.000 lavoratori irregolari nel nostro Paese e credo che una stima effettuata oggi ci porterebbe a risultati non molto diversi circa le dimensioni dell'irregolarità. Come sapete, questo è un fenomeno molto diffuso e le cause della diffusione dell'irregolarità sono naturalmente molteplici, ma una delle più forti è l'alto livello di economia sommersa: il nostro Paese ha quasi un quinto del proprio PIL che deriva da attività non alla luce del sole e una quota di lavoro irregolare che è superiore a quella del PIL generato dal sommerso. Questo è, naturalmente, un quadro di riferimento preoccupante. In questo quadro di irregolarità e di economia sommersa, ci sono delle punte di fattispecie di gravissimo sfruttamento del lavoro nel territorio, sia nella fase del reclutamento, sia nella fase dell'intermediazione, sia nella fase dell'impiego dei lavoratori. Naturalmente, l'alto livello di sfruttamento genera non solo danni ovvii per l'integrità del lavoratore stesso, ma genera economia al nero, distorce il mercato, distorce la concorrenza, quindi è un fattore di disturbo gravissimo del nostro sistema produttivo e del nostro sistema sociale. Aggiungo, ancora, che gran parte delle informazioni a nostra disposizione ci danno risultanze preoccupanti circa la diffusione del grave sfruttamento; il grave sfruttamento e il fenomeno di caporalato a questo connesso è diffuso in quasi tutte le nostre Regioni, anche se ha delle punte in particolari Regioni, che tutti conosciamo. Riguarda molte etnie di immigrati, non una sola ma gran parte di esse. Riguarda molte attività produttive: non solo quelle stagionali della raccolta dell'uva o del o del pomodoro, ma anche attività manifatturiere come nel settore tessile; attività di costruzione nel settore edile e varie aree del settore dei servizi. Quindi, c'è un diffuso sistema di intermediazione La gran parte dei clandestini sbarcati a Lampedusa racconta di avere un referente in Italia e questo referente in molti casi è quello quello che definiremmo un caporale, cioè un intermediatore abusivo di manodopera. Allora, l'obiettivo primo della legge è naturalmente quello di contrastare le forme più gravi di sfruttamento del lavoro, proteggendone le vittime, e di rafforzare il regime sanzionatorio per la somministrazione e l'impiego del lavoro irregolare. Ricordo che la tolleranza che c'è nel nostro Paese per queste forme gravissime di sfruttamento crea anche una insensibilità generalizzata di fronte

finiamo per non accorgerci nemmeno della gravità del fenomeno del lavoro irregolare, che consideriamo un fatto normale. Questo è un risultato davvero grave della situazione. Quindi, oltre alla protezione delle vittime del grave sfruttamento, questo provvedimento cerca anche cerca anche di prosciugare, ridurre, circoscrivere l'economia sommersa, che è la causa maggiore dell'irregolarità del caporalato e del grave sfruttamento. I contenuti sono dettagliati nella relazione. Si introduce un reato di grave sfruttamento che si riferisce al reclutamento di lavoratori o all'impiego di lavoratori che vengono sottoposti a grave sfruttamento mediante violenza o minaccia o mediante intimidazioni o che pure esercitano il lavoro in forme degradanti.

la non inclusione delle famiglie che non esercitano impresa qualora il numero degli irregolari al lavoro nella famiglia non superi il numero di due. Abbiamo qui voluto eliminare una fattispecie molto diffusa di irregolarità che è quella delle assistenti familiari sia nella cura dei bambini che degli anziani, per non mettere a rischio una fetta davvero consistente della popolazione. Infine, si introduce una nuova fattispecie delittuosa per l'utilizzo di stranieri irregolarmente soggiornanti qualora questo utilizzo sia avvenuto attraverso l'intermediazione abusiva di manodopera. Questa è la struttura della Questa è la struttura della normativa che qui si propone, che ho cercato di mettere in un contesto più generale e mi auguro che anche in Aula si possano raggiungere quelle ampie convergenze che si sono raggiunte in Commissione.

Signor Presidente, il disegno di legge di cui l'Aula del Senato inizia l'esame dimostra come sia possibile e necessario adeguare la legislazione con misure dirette e condivise, anticipando una revisione generale e radicale della normativa in materia di immigrazione. L'esame presso le Commissioni affari costituzionali e lavoro ha prodotto un testo che, seppur parzialmente diverso da quello originario del disegno di legge, il quale già definiva una casistica rigorosa delle forme possibili di sfruttamento sul lavoro, assicura comunque garanzie necessarie a chi intenda denunciare i casi di grave sfruttamento consentendo di punire i responsabili. Tale obiettivo è stato raggiunto anche grazie alle modificazioni apportate nel comune lavoro dei Gruppi nelle Commissioni riunite; tuttavia va preliminarmente ribadito l'apprezzamento per l'iniziativa governativa che aveva il pregio di definire un elenco dettagliato di situazioni di grave sfruttamento del lavoro, in modo tale da evitare possibili difformità interpretative in ordine a comportamenti penalmente rilevanti. Peraltro, la fattispecie delittuosa in questione riguarda non solo i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma anche quelli con regolare permesso di soggiorno, nonché gli stessi lavoratori italiani spesso sottoposti a situazioni di sfruttamento. L'introduzione di più incisive misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera, particolarmente accentuato verso i lavoratori extracomunitari irregolari, consente di dare una prima risposta ad un problema che è diffuso in ogni settore produttivo (in particolare in quelli dell'edilizia e dell'agricoltura, ove risulta maggiormente radicato). Proprio la condizione di clandestinità in cui sono costretti a trovarsi questi lavoratori per via di una normativa sull'immigrazione assurdamente punitiva e contraria agli stessi interessi economici dei settori produttivi, li induce a dover subire silenziosamente condizioni intollerabili di sfruttamento, condizioni che hanno raggiunto livelli tali da non potere dire garantiti i diritti fondamentali delle persone. Per questo l'originaria modifica all'articolo 18 del testo unico dell'immigrazione, nel prevedere che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale fosse applicabile anche in presenza di una situazione di «grave sfruttamento del lavoro», elencava una serie di condizioni che qualificavano tale condizione. Possiamo citare la previsione di una retribuzione particolarmente ridotta anche rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria; la reiterazione di violazioni della disciplina vigente in tema di orario di lavoro, di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (con la conseguente esposizione dei lavoratori a gravissimi pericoli), fino ai casi di reclutamento ai limiti della tratta in schiavitù (il ben noto fenomeno del caporalato). Poiché però il fenomeno non interessa unicamente la manodopera extracomunitaria, si è addivenuti ad un testo più ampio, che intende colpire le forme più gravi di sfruttamento anche per quanto riguarda i lavoratori italiani. Per quanto concerne i lavoratori extracomunitari si raggiunge ugualmente l'obiettivo di garantire il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, previsto dall'articolo 18, comma 1, del testo unico, attraverso l'inclusione del grave sfruttamento della manodopera nei casi per i quali si ha l'arresto in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale. Il testo originario aveva suscitato alcune perplessità, in primo luogo per l'esclusione dello straniero vittima di grave sfruttamento dai programmi di assistenza e integrazione sociale,

ed era stata sottolineata la necessità di chiarire, se per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in presenza di una situazione di grave sfruttamento del lavoro, previsto con una novella all'articolo 18 dello stesso decreto legislativo, fosse comunque richiesta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 di quello stesso articolo, con particolare riferimento a quello dell'attualità di un pericolo incombente per l'incolumità del lavoratore. L'introduzione della fattispecie penale di grave sfruttamento dell'attività lavorativa tra le ipotesi di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, che disciplina i casi di arresto in flagranza di reato, costituisce dunque il presupposto per l'applicazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione. La necessità di un intervento è comunque indubitabile. La presenza sul territorio nazionale di veri e propri schiavi, sfruttati e sottopagati, alloggiati in luridi tuguri e massacrati di botte se protestano, è una realtà intollerabile per un Paese civile. Una realtà che, se teoricamente riguarda tutti i lavoratori, sappiamo comunque che interessa soprattutto migranti, regolari e non, rifugiati e asilanti. E tanto più coloro che, spesso minori, sono costretti ad una situazione di clandestinità da una normativa, come la legge Bossi-Fini, che è talmente punitiva e vessatoria da indurre i migranti a tentare la via illegale per l'ingresso nel nostro Paese. I clandestini sono, per la loro stessa condizione, fatalmente esposti alla violenza ed allo sfruttamento lavorativo ad opera di imprenditori senza scrupoli. Si tratta di piccole aziende che, quando devono assumere personale stagionale per la raccolta nei campi, scelgono la «scorciatoia» del caporalato, o di grandi imprese che sono consapevoli dei subappalti che impiegano l'immigrazione clandestina. Il fenomeno riguarda diversi territori, come è già stato dettagliatamente denunciato dalle associazioni umanitarie e dai sindacati, che hanno documentato le inaccettabili condizioni igieniche e lavorative degli sfruttati. Il 40 per cento di queste persone vive in edifici abbandonati; il 36 per cento vive in spazi sovraffollati; più del 50 per cento non dispone di acqua corrente; il 30 per cento non ha elettricità; il 43,2 per cento non dispone di *toilette*; la maggior parte riesce a mangiare solo una volta al giorno e spesso si nutre dello stesso prodotto di raccolta, con enormi limiti nell'apporto calorico e nutrizionale. In conseguenza di tutto ciò le patologie riscontrate sono spesso gravi. In queste condizioni di lavoro e di vita si vengono a trovare non solo immigrati irregolari (51,4 ma anche rifugiati (6,3 per cento), richiedenti asilo (23,4 per cento) e persone con permesso di soggiorno (18,9 per cento). Le stesse condizioni di sfruttamento e precarietà riguardano anche cittadini italiani, come è dimostrato dalle quotidiane notizie di cronaca sulle tante «morti bianche» di donne, minori e uomini ridotti in schiavitù a lavorare in turni massacranti e senza alcuna protezione. È quindi un dovere contrastare attivamente i fenomeni di grave sfruttamento della manodopera, del caporalato e dello schiavismo, assicurando alla magistratura e alle forze di polizia, agli enti locali, alle organizzazioni professionali dei produttori, dei coltivatori e dei consumatori, alle organizzazioni sindacali e agli ispettori del lavoro, norme adeguate ed efficaci, tra le quali rientra anche il codice penale. Si tratterà poi di controllare la filiera produttiva e di trasformazione dei prodotti agroalimentari, il settore tessile piuttosto che quello edilizio o manufatturiero, in modo che gli operatori senza scrupoli non danneggino i concorrenti azzerando le tutele sociali e i diritti della persona sul luogo di lavoro. Fondamentale rimane però il sostegno alle vittime dello sfruttamento che denunciano violazioni alle leggi dello Stato e ai diritti umani, dando piena attuazione, a tale fine, all'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'immigrazione, che prevede l'accesso alla protezione per la collaborazione di giustizia a tutti i migranti che denunciano tali situazioni di sfruttamento e schiavismo, indipendentemente dal loro *status* di presenza sul territorio italiano. Auspichiamo quindi che, anche apportando qualche miglioramento attraverso opportuni emendamenti, si approvi questo testo in vista di un recupero dell'originario spirito del disegno di legge governativo attraverso una profonda e generale riforma del testo unico sull'immigrazione, da avviare rapidamente all'esame delle Camere. Occorre, infatti, colpire le strategie che portano alla precarizzazione sistematica del lavoro migrante che, attraverso un meccanismo a polmone, viene attirato o espulso a seconda delle esigenze dei datori di lavoro. Queste politiche di rotazione-precarizzazione sono state caratterizzate da: espulsione amministrativa come meccanismo di regolazione del mercato del lavoro; clandestinizzazione dell'immigrazione con conseguente «normalizzazione» della precarietà; differenziazione gerarchica tra gli immigrati in base alla provenienza e alle presunte affinità etniche; selezione della manodopera migrante nei Paesi di origine o all'atto dell'entrata nel nostro Paese. L'attuale normativa sull'immigrazione è pensata dunque per soddisfare esplicitamente queste condizioni di sfruttamento, rifiutando di vedere il migrante come soggetto sociale e considerandolo soltanto come pura forza-lavoro.

Voglio, però, integrare con alcune osservazioni che mi paiono necessarie rispetto a questo provvedimento ma più in generale a tutto il tema. Le considerazioni sono di tre ordini di fattori. In primo luogo, è vero che esiste questo fenomeno, diffuso in alcune Regioni, ma non credo in modo particolare in alcune Regioni o in alcune stagioni perché io, pur venendo dal Nord, vedo come in alcuni settori, ma anche nelle case, nei rapporti con le cosiddette badanti, spesso si determinano situazioni che potrebbero essere definite anche

colui che definiamo sfruttatore in generale e colui che qui definiamo sfruttato, e dovremmo chiederci il perché ci sia questa connivenza nel mantenere un regime di illegalità che dovrebbe essere sconveniente per entrambe le parti. Spesso accade, Presidente, che chi viene da altri Paesi, e magari si trova in condizione di irregolarità

preferisce egli stesso non fare un contratto regolare, perché questo gli comporterebbe un certo reddito monetizzato e una quota parte contributiva-previdenziale che non vede; preferisce invece monetizzare tutto

Ciascuno di noi conoscerà situazioni di questo genere, come quella per cui badanti che vengono magari da Paesi entrati di recente nell'Unione Europea o da altri Paesi al di fuori dell'Unione vogliono essere tenute in nero e magari utilizzano il meccanismo del soggiorno temporaneo di tre mesi, interrompendolo per un periodo di tre mesi e alternandosi con altre persone (magari in due persone coprono un intero anno a turni di tre mesi ciascuna). In questo modo riescono a monetizzare di più e ad avere redditi maggiori. Questa è una delle situazioni. Seconda considerazione:

è assolutamente competitivo rispetto al lavoro irregolare, con distanze che possono essere abissali. Per cui, se dovessimo impiegare lavoratori totalmente regolarizzati in alcune attività probabilmente il costo del prodotto finale sarebbe elevatissimo. Facciamo un esempio banale e storico, quello del pomodoro. Nel settore della raccolta del pomodoro registriamo una vastissima irregolarità e un'immigrazione temporanea di persone che lavorano totalmente al nero; questa è l'unica leva economica per cui il nostro pomodoro riesce ancora un po' a competere con quello cinese. Dobbiamo allora trovare un accordo, o meglio, una soluzione nell'organizzazione della nostra economia. O noi sbarriamo la strada al pomodoro cinese

sempre fare i conti con livelli di irregolarità e di estraneità alla legge, perché ne produrremo noi, attraverso le nostre norme, le premesse assolutamente obbligatorie. rassegniamoci al fatto che non si coltivi più pomodoro. È una scelta, non so quale sia la migliore ma certo il problema dobbiamo porcelo in termini più generali; non dobbiamo semplicemente lavare la nostra coscienza dicendo che abbiamo previsto una sanzione penale grave per chi sfrutta il lavoro e che adesso tutto è a posto. Terza considerazione: questo provvedimento, al quale, ripeto, guardo con favore, si inscrive più in generale nella politica dell'immigrazione.

È giusta la severità con chi sfrutta il lavoro, indipendentemente dalla carta d'identità di chi viene sfruttato ed è giusto avere maggiore rigore laddove le condizioni contrattuali siano più deboli (in questo caso parliamo di extracomunitari); è giusto anche introdurre un incentivo a sfuggire all'irregolarità, come la concessione per fini sociali del permesso di soggiorno;

Tutte le norme contenute nel disegno di legge Amato-Ferrero che, aprendo le maglie all'ingresso, favoriscono la permanenza in assenza di lavoro, favoriscono obiettivamente anche il caporalato,

manifestiamo sentimenti di buona accoglienza nei confronti di tutti, se qualcuno non ha lavoro lo manteniamo e decidiamo che può rimanere sul territorio, magari anche per un anno, in cerca di nuovo lavoro, sanzioniamo penalmente il caporalato, per poi accorgerci che il caporalato fa agio proprio su quella

buone letture; abbiamo fatto buone scuole, grazie a Dio). Credo che questo provvedimento di per sé

così elevate. Quanto più è conveniente il sommerso, infatti, tanto più vi si farà ricorso e tanto più inutile sarà la sanzione penale. È lo stesso discorso che vale per l'evasione fiscale.

la legge Bossi-Fini contenga manchevolezze, perché, per esempio, prevede che gli ingressi siano basati sull'ordine in cui si presenta la domanda. Sono dell'opinione che, invece, bisogna selezionare gli ingressi in base alle competenze specifiche. Dobbiamo cominciare a ragionare come si fa in tutta Europa, dove si seleziona la manodopera in base sulla sua qualificazione e si fanno entrare dall'esterno dell'Unione Europea le persone in base alle loro capacità

Signor Presidente, desidero sollecitare alcuni atti di sindacato ispettivo

per la dismissione da parte del demanio militare del Forte Appio e il suo passaggio al patrimonio archeologico del Parco dell'Appia antica; "Il link apre una nuova finestra"), presentata il 2 maggio al Ministro dell'ambiente e a quello dell'interno sulle discariche abusive di rifiuti tossici e nocivi nel Comune di Giugliano in Campania. Mi rivolgo alla benigna attenzione della Presidenza del Senato per ottenere risposta dal Governo.